dalla Commissione per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione «La Commissione programmazione economica, bilancio, tenuto conto dei nuovi chiarimenti forniti dal Governo e a rettifica del parere reso il 2 marzo scorso, esaminato il testo in titolo, esprime parere non ostativo nel presupposto che le attività di coordinamento connesse all'attuazione delle squadre investigative comuni, già in essere, siano realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che l'espletamento di funzioni di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti distaccati, ovvero ai rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, non dia luogo al riconoscimento di indennità aggiuntive ed infine che sia garantita, da accordi esistenti, la reciprocità per i danni causati dal funzionario straniero o distaccato nello svolgimento dell'attività di squadra investigativa comune. In relazione agli emendamenti, esprime parere di nulla osta sulle proposte 2.100. 2.101 e 4.102 negli identici presupposti del parere di nulla osta reso sul testo. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.103 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.100. Il parere è altresì favorevole su tutti i restanti emendamenti».

modificando l'emendamento del Governo in tal senso: «Il capo della squadra, da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria». nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria». Vi sono infatti alcuni che non sono ufficiali nelle forze di polizia.

offerta a quest'Assemblea dal relatore, senatore D'Ambrosio, sia nel corso della discussione generale. Si tratta di uno strumento di snellimento delle procedure procedure richiesto da molti Paesi: ora anche l'Italia si dota di questo strumento importante, in particolare nel contrasto ai crimini transnazionali, e quindi con un sostanziale superamento della burocrazia delle rogatorie attraverso la snellezza della squadra investigativa sovranazionale composta

L'Unione europea ha poi disciplinato le squadre, dapprima con la Convenzione di Bruxelles del 2000 e quindi con successiva decisione quadro del Consiglio del 2002. Sono seguiti negli anni accordi e convenzioni: penso a quella dell'ONU contro la corruzione e all'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra Unione europea e Stati Uniti.

Ormai da tanti anni la criminalità organizzata travalica i confini dello Stato, cooperando a livello internazionale per gestire mercati comuni come quello delle armi, della droga come quello delle armi, della droga e della tratta di esseri umani. La pericolosità di gruppi criminali si è moltiplicata a seguito del recente allargamento della comunità europea e della conseguente Siamo inoltre di fronte a un numero sempre crescente di aree di crisi in cui la criminalità organizzata internazionale gioca un proprio

nella sua relazione ha illustrato perfettamente la decisione quadro del Consiglio europeo del giugno 2002 su cui si fonda questo provvedimento). Le squadre investigative comuni sono indubbiamente uno strumento operativo di estrema importanza, da utilizzare in materia di contrasto alla criminalità organizzata

Questo disegno di legge va proprio nella direzione di rafforzare la cooperazione investigativa tra le forze di polizia che contrastano questi gravi reati di criminalità organizzata,

Questo strumento può diventare, se lo vorranno le procure, un potente strumento di contrasto dell'immigrazione clandestina, del traffico di clandestini via mare proveniente dalle coste nordafricane, in particolare da Tunisia e Libia. Ma presupposto indispensabile per una efficace cooperazione investigativa transnazionale è l'avvio di indagini interne su questi gravissimi reati che si consumano quotidianamente sotto i nostri occhi senza che un procuratore competente, in particolar modo della Sicilia, senta il bisogno di avviare almeno un'indagine per il reato di tratta di esseri umani o per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, presenteremo un'interrogazione per avere i dati in merito alle indagini avviate dai procuratori della Repubblica su queste due fattispecie di reato. Questo strumento di cooperazione investigativa può - ripeto - agevolare le indagini transnazionali su questi gravi reati, ma occorre che almeno un procuratore della Repubblica,un nostro Le forme di cooperazione fra i gruppi criminali di nazionalità diverse finalizzate alla gestione del mercato criminale del traffico di clandestini via mare devono essere affrontate con una nuova cooperazione investigativa sovranazionale. Di fronte a queste nuove sinergie criminali internazionali deve essere contrapposta una risposta investigativa unitaria e sovranazionale. Questo disegno di legge nasce proprio a questo scopo,

ricordo che quel Patto europeo, fortemente voluto a suo tempo dalla Francia, recita testualmente: «Gli Stati membri che si trovano a dover affrontare flussi di migranti massicci e sproporzionati rispetto alla propria capacità di accoglienza devono poter contare sull'effettiva solidarietà degli altri Stati membri». La solidarietà tra Stati europei deve essere dunque ancora più forte, e questo disegno di legge la rafforza nel settore della cooperazione investigativa.

e anche perché si tratta di un provvedimento che nell'Aula del Senato ha già avuto occasione di verifica, di confronto, di discussione e di voto. tratta infatti di un'iniziativa parlamentare che precede l'attuale legislatura; ciò indica un lungo percorso di attenzione e di convergenza da parte delle forze politiche e dei Gruppi. Sicché, nel motivare il voto

già con il Trattato di Prüm sono state messe in atto importanti collaborazioni al fine della repressione dei reati più gravi, quelli appunto collegati alla criminalità organizzata e, tra l'altro, ci si è dotati di una banca dati del DNA che potrà consentire con estrema velocità e certezza l'identificazione delle persone che commetteranno reati. Queste ed altre motivazioni sono a supportare il voto favorevole su un provvedimento che, è vero, forse arriva tardivamente, ma arriva in maniera condivisa, ed è quindi importante che questo segnale sia sia espresso oggi dal Senato e dal Parlamento.

cui, nella lotta fra la criminalità organizzata e chi deve combatterla, c'è la necessità di agire immediatamente.

a tutti quei reati che possono interessare comunque più Stati. Finalmente, qualora più Stati si occupino di una stessa indagine, potranno stabilirsi rapporti diretti e immediati tra i rispettivi magistrati, oltreché tra le polizie giudiziarie, tra cui già esiste questa collaborazione. Questo, naturalmente, consentirà di combattere in maniera estremamente più efficace la criminalità organizzata e di ottenere conseguentemente successi veramente definitivi.

È da svariato tempo che la criminalità organizzata opera in modo transnazionale. I traffici si articolano tra Paesi non solo situati all'interno dell'Unione europea, ma anche fuori, con postazioni e basi che la stessa criminalità organizzata italiana spesso ha realizzato in Paesi esterni all'Unione europea, produttori, ad esempio, di droga. E allora, la possibilità che, attraverso accordi tra Stati e attraverso l'attuazione dei principi affermati dal Consiglio europeo, si possa arrivare ad una collaborazione fattiva sul versante delle indagini è un importante passo avanti. Ci dobbiamo però dire chiaramente una cosa. C'è una sovrastruttura complessiva magistrati di collegamento, Eurojust, Europol, magistrati appartenenti alla rete giudiziaria, oggi squadre investigative - che va certamente semplificata.

in grado di interagire con particolare efficacia, la lotta al crimine transnazionale sarà sempre segnata da estrema difficoltà.

fine e al traguardo di un percorso iniziato già da svariati anni. Mi riferisco ad una legislazione europea omogenea sul versante del diritto sostanziale, ma anche su quello del diritto processuale,

nello scambio di notizie e nella collaborazione. Insomma, una serie di strumenti veramente efficaci per contrastare un crimine sempre più potente e più forte che opera rapidamente in vari Paesi e che inonda i Paesi dell'Unione europea con denaro sporco riciclato da traffici illeciti sempre più lucrosi. Il voto del mio Gruppo sarà quindi favorevole. Salutiamo -

e vista l'unanimità della Commissione igiene e sanità. Vorrei anzitutto spendere qualche parola sulla patologia diabetica, che è stata definita una malattia sociale proprio per la sua eccezionale diffusione. Si stima infatti che quattro milioni di italiani adulti soffrano di tale malattia; anche il diabete infantile è purtroppo molto diffuso: sono più di 20.000 i bambini e i ragazzi fino a 14 anni affetti da tale patologia. Il dato allarmante è che questo bilancio è destinato ad aumentare:

Vorrei mettere in luce la sofferenza silenziosa che vivono queste persone, e in ultimo, ma non per importanza, ricordare i costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a sostegno di tali pazienti, che ammontano al 9 per cento della spesa sanitaria totale. In cifre, lo Stato spende 9,22 milioni di euro l'anno: una somma consistente e significativa, soprattutto se si considera che il 75 per cento di questa spesa è utilizzato per curare le complicanze. Fortunatamente, in Italia esistono 120 120 centri di diabetologia, che garantiscono la diagnosi, la presa in carico e l'accompagnamento delle persone diabetiche: ci appelliamo al Ministro affinché possano continuare a lavorare con professionalità e disponibilità. destinano le loro risorse umane ed economiche ad affrontare le complicanze, ma è auspicabile - grazie ad un migliore e maggiore autocontrollo - che l'attività preziosa e insostituibile svolgono non sia più dedicata in prevalenza alla gestione delle complicanze. Dai dati che vi ho appena illustrato, emerge con lampante evidenza la necessità di attuare una politica di prevenzione del diabete, che non solo migliorerebbe le condizioni di salute dei pazienti, ma comporterebbe anche un significativo contenimento della spesa pubblica,

di cui siamo primi firmatari io ed il Presidente della 12ª Commissione igiene e sanità, il senatore Antonio Tomassini. Si tratta di una mozione dal contenuto e dagli effetti importanti, supportata da un sostegno trasversale, a dimostrazione del fatto che, quando si parla di prevenzione di una malattia cronica, si dimenticano i colori politici e si ha a cuore la salute dei cittadini. La mozione trae origine da un'osservazione empirica del mondo diabetico. Com'è a tutti noto, il Servizio sanitario nazionale garantisce al paziente, oltre alla diagnosi ed alla cura, anche la somministrazione di tutti i presidi diagnostici necessari alla terapia vitale. In concreto, il paziente può reperire i presidi o presso i centri di diabetologia di aziende sanitarie o di ospedali oppure rivolgendosi alle farmacie: purtroppo, però, è fondamentale ricordare che la distribuzione dei presidi non è uguale su tutto il territorio nazionale. Gli importi che il Servizio sanitario eroga per effettuare il rimborso dei presìdi diabetici variano da Regione a Regione: solo per citare il minimo ed il massimo che risulta dai dati in nostro possesso, ricordo per esempio che in Veneto il prezzo unitario rimborsato per ogni striscia reattiva di rilevazione della glicemia

ad un massimo di 0,85 euro, ossia più del doppio: ciò sta a significare che a carico del bilancio dello Stato gravano costi di diverso importo a seconda della Regione di riferimento, sebbene in pratica vengano erogati presidi identici e comparabili. L'altro dato importante da cui muove la mozione è la constatazione che oggi in Italia solo il 60 per cento delle persone diabetiche pratica l'autocontrollo,

Un costante controllo glicemico consente le modifiche terapeutiche che favoriscono condizioni di vita migliori per le persone diabetiche e una minore probabilità di insorgenza delle complicanze. Le complicanze insorgono anche per una predisposizione del fisico della persona diabetica. Però, l'autocontrollo ed una corretta terapia facilitano sicuramente l'insorgenza in tempi più lontani oppure la non insorgenza delle complicanze. I frequenti ricoveri ospedalieri limitano il benessere vitale e la regolare attività professionale del soggetto diabetico, causando anche danni all'intera economia, e ovviamente al servizio Sanitario nazionale. Oggi vorrei anche sottoporre alla vostra attenzione due fatti allarmanti che devono suscitare il nostro unanime sconcerto, richiamandoci tutti ad un atto di responsabilità. In passato alcune aziende sanitarie avevano indetto delle gare pubbliche per la fornitura di presidi diabetici adottando l'unico criterio del prezzo più basso, senza considerare le indicazioni provenienti dai diabetologi e prescindendo dalla valutazione del quadro clinico e dello stile di vita di ogni singolo paziente. Fortunatamente quelle gare sono state revocate giusto in tempo. La stessa cosa però non è avvenuta quando sono stati immessi nel mercato dispositivi privi degli essenziali requisiti di qualità e che rilevavano in maniera errata il tasso di glicemia nel sangue. Questo è avvenuto a Napoli, nella Regione Campania. Dispositivi che solo dopo continui ricorsi al pronto soccorso sono stati ritirati per evitare ulteriori gravi danni ai pazienti diabetici. Questi errori non possono e non devono più accadere, perché in gioco ci sono delle vite umane. Bisogna dunque agire d'anticipo e predisporre una concreta strategia di prevenzione che garantisca al paziente diabetico uniformità di cure a livello nazionale. Per fare ciò, ad oggi manca un tassello importante, signor Ministro: l'inserimento dell'autocontrollo nei livelli essenziali di assistenza. È un obiettivo che ci diamo, non oggi ma nel medio periodo. Speriamo che questo obiettivo sia realizzato, perché risponde non solo ad un criterio di condizioni migliori di vita per le persone diabetiche, ma anche ad un obiettivo corretto dal punto di vista scientifico della diabetologia oggi più illuminata, e anche a un obiettivo corretto dal punto di vista economico. Questa sarebbe la vera soluzione per attuare una concreta prevenzione della malattia diabetica. Nella speranza che questo avvenga in tempi rapidi, noi chiediamo l'impegno del Governo a promuovere una corretta diagnosi e terapia di tutte le patologie croniche (di tutte le patologie croniche, e del diabete *in primis*)*,* e ad ammettere i cittadini all'utilizzo di una pluralità di dispositivi medici che siano conformi ai requisiti della normativa comunitaria e alle innovazioni tecnico-scientifiche e rispondano alle esigenze cliniche e personali del paziente. Sembra una richiesta normale e naturale. possiamo quasi ritenere assurdo di dovercene occupare oggi in Aula. Ma siccome la realtà prevede una pluralità di situazioni e di condizioni all'interno del nostro Paese, è doveroso che noi oggi ce ne occupiamo. Siamo costretti a farlo perché finalmente si ponga fine a questo assurdo modo di operare che caratterizza una parte del Servizio sanitario nazionale. Il nostro dovere inderogabile previsto dalla Costituzione è di prendere in carico coloro che si curano in modo non adeguato, coloro che non effettuano l'autocontrollo e coloro che ancora oggi ignorano di essere diabetici (ce ne sono ancora molti). Si chiede in modo chiaro e semplice un impegno concreto affinché vengano predisposte linee guida che individuino precisi parametri di riferimento per la fornitura dei presidi per diabetici, che costituiscono strumenti essenziali per il paziente diabetico

ipoglicemizzanti. Lo scopo finale è quello di garantire la qualità dei dispositivi, la libera scelta del paziente, un'uniformità su tutto il territorio nazionale e, finalmente, un risparmio della spesa pubblica. Ringrazio in modo particolare tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione e ringrazio anche il Ministro perché ha collaborato con noi affinché questa mozione venisse calendarizzata e approvata all'unanimità.

a livello mondiale, che aggredisce la salute umana in maniera silente, sia oggi un'emergenza clinica, sociale ed economica e non solo un problema di ordine sanitario.

una rivoluzione di ordine culturale. Questa è la tipica malattia, signor Ministro, che si affronta con l'unione tra territori e ospedali,

nella salvaguardia assoluta dell'autonomia regionale, deve essere quello di curare soprattutto i deboli e di servire i cittadini. Pertanto, quando qualche autorità periferica

sociosanitaria, signor Ministro, perché non pensare anche a un aiuto alle famiglie? Saranno tutti fondi che serviranno per abbattere questa cifra astronomica che il Servizio sanitario nazionale spende. oltre all'impegno alla ricerca, signor Ministro, perché non aiutare le associazioni, che svolgono un ruolo importantissimo? Ho vissuto esperienze incredibili con associazioni di alcune Regioni che funzionano egregiamente

Ripeto, abbiamo accertato che non era stato così: la guardia medica ha dichiarato la sua incompetenza addirittura di fronte a cittadini che non erano nati in Veneto. Credo che tale episodio

Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Centro di formazione professionale «ENAIP» di Tione di Trento, ai quali rivolgo il nostro benvenuto e un augurio per la loro attività scolastica.

Ministro, ho condiviso e firmato la mozione di cui è prima firmataria la senatrice Baio. Il diabete è una malattia di grande rilievo sociale ed esercita un notevole impatto sulla salute pubblica per l'entità della sua diffusione e per la gravità delle sue complicanze. La stima della prevalenza del diabete nella popolazione italiana si aggirerebbe attorno al 4,5-4,7 per cento, con previsione del raggiungimento del 10 per cento Un'approfondita ricerca sulla spesa per la cura della patologia diabetica e delle sue complicanze condotta in 8 Paesi d'Europa (progetto CODE-2) indica che il diabete richiede cospicue risorse, soprattutto quando è causa di complicanze. In Italia assorbe il 6,65 per cento della spesa sanitaria complessiva. A titolo di esempio, in una realtà aziendale della Regione Piemonte il costo per la sola fornitura di materiale a pazienti diabetici (con esclusione, quindi, dei costi indiretti derivanti dalle complicanze) si è attestato nel 2010 sulla cifra di oltre 3,8 milioni di euro, il che significa che ogni cittadino di quell'ASL (diabetico o no) ha sopportato una spesa *pro capite* di circa 11,5 euro l'anno. A questi costi, direttamente incidenti sul Fondo sanitario nazionale, occorre aggiungere quelli derivanti dalle assenze dal lavoro dei pazienti e quelli legati ai prepensionamenti degli stessi per invalidità.

Ben si comprende, quindi, la notevole rilevanza che il fenomeno assume sia per l'impatto sulla salute delle singole persone, sia per la notevole entità delle risorse economiche coinvolte. con riferimento alla salute dei singoli appare prioritaria una scelta improntata alla prevenzione del fenomeno attraverso campagne di formazione ed informazione che coinvolgano tutti i soggetti istituzionali (tra cui, sanità e scuole) ed associazioni (soprattutto quelle di volontariato). La sensibilizzazione delle persone diabetiche sull'importanza dell'autocontrollo poi consentirebbe non solo una maggior consapevolezza di sé e del proprio stato di salute, ma anche un migliore e più efficace utilizzo delle risorse messe a disposizione, contribuendo a limitare il più possibile il deprecabile fenomeno degli sprechi. In questo ambito appare fondamentale la collaborazione tra i medici specialisti diabetologi ed i medici di medicina generale. Dal punto di vista più strettamente economico, il fenomeno relativo alle ASL che indicono gare pubbliche per la fornitura di presìdi per soggetti diabetici (strisce e lancette) adottando come unico criterio quello del prezzo più basso ha immediata ripercussione sulla qualità del prodotto fornito e, di conseguenza, sulla qualità dell'assistenza erogata. Importante, allora, appare la necessità di regolamentare le modalità di distribuzione optando per questa soluzione che appare economicamente più vantaggiosa, salvaguardando sempre e comunque la qualità del prodotto. In Piemonte il rimborso regionale alle farmacie avviene sulla base di 0,65 euro, mentre il costo derivante dalla distribuzione diretta da parte delle ASL si fermerebbe a 0,44 euro, con un risparmio di circa un terzo. potrebbe diventare un percorso da intraprendere. Un miglior utilizzo delle risorse economiche a disposizione garantirebbe la sostenibilità del sistema di interventi a favore dei soggetti diabetici: non si tratta solo di spendere meno per risparmiare, ma di spendere bene per permettere il medesimo accesso alle cure, in modo uniforme su tutto il territorio, perché ad oggi ancora così non è.

ancora una volta questa Assemblea, dopo la mozione approvata nel 2009 con un protocollo di intesa, impegno proseguito nel 2010 con l'Osservatorio,

Dobbiamo ricordarci che si stimano 19.000 persone ogni giorno nel mondo che svilupperanno il diabete nei prossimi 20 anni.

(testo 2) affronta un problema collettivo estremamente importante e diffuso, soprattutto in relazione alla cura di tale malattia. La cura appropriata del diabete, oltre a permettere una buona qualità di vita ai pazienti,

neuropatico, o oculare. Purtroppo nell'ambito delle diverse Regioni, e anche all'interno di uno stesso territorio regionale, i presìdi vitali per il paziente diabetico sono erogati con diverse modalità e secondo differenti importi di rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale. Questa mozione tende a sottolineare la disomogeneità sostanziale di rimborsabilità: non è accettabile che nel Lazio il prezzo unitario rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per ogni striscia reattiva di rilevazione della glicemia sia pari a 0,81 euro, a fronte di un rimborso di 0,513 euro praticato in Lombardia (in tale ultima Regione, tale rimborso si riduce a 0,125 euro nel distretto di competenza dell'ospedale civile di Brescia).

a promuovere una corretta informazione, diagnosi e terapia di questa patologia cronica; a erogare una pluralità di dispositivi medici che siano conformi ai requisiti e alle innovazioni tecnico-scientifiche e rispondano alle esigenze cliniche e personali dei pazienti; a predisporre un sistema di certificazione di qualità delle imprese che intendano concorrere alla fornitura dei presidi;

Signor Ministro, per rendere utile questa discussione odierna mi consenta però alcune considerazioni.

della sanità è cosa ben diversa dalla politica di tutela della salute. In questa mozione lei avrà notato che si fa riferimento a situazioni di appalti per l'acquisizione di presidi diagnostici e terapeutici della cura del diabete che non rispondono a criteri di sicurezza, di efficienza, di qualità nella risposta delle prestazioni, sentore del fatto che spesso in molte ASL del nostro Paese i direttori generali sono più orientati dal pareggio dei conti e quindi a fare appalti al massimo ribasso, per la massima economia piuttosto che a porre quell'attenzione necessaria a far sì che i presidi diagnostici e terapeutici siano veramente funzionali alla cura dei pazienti. Tra l'altro, poiché provengo dalla Regione Abruzzo, in questi mesi, all'insegna del piano di rientro, sono stati eliminati i sussidi economici per aiutare i pazienti oncologici, anche in fase terminale. ci rendiamo conto che spesso si vedono due realtà diverse: una del Parlamento in cui si manifesta una grande condivisione e un'altra, frastagliata a livello regionale, in cui in realtà le situazioni sono ben diverse.

che un'adeguata prevenzione per la salute fa risparmiare molto di più di quello che si possa pensare e soprattutto, pur non ottenendo effetti diretti e immediati, i risparmi si vedono nel corso del tempo.

per quasi il 6,6 per cento sul Fondo sanitario nazionale. Però lei sa, signor Ministro, che questa percentuale diventa tre, quattro o anche cinque volte tanto se si vanno a curare quelle patologie e complicanze microvascolari e cerebrovascolari di cui il diabete è

I contenuti della mozione non fanno altro che richiamare quelli della legge n. 115 del 1987, una legge quadro che già affrontava

attraversato 12-13 anni, trova ancora difficoltà nella sua applicazione. I principi cardine di questa legge quadro, signor Ministro, erano due. dire la necessità di uniformare i trattamenti sul piano dei modelli organizzativi e dei criteri diagnostici e terapeutici in tutte le Regioni.

ma nel nostro Paese abbiamo qualche difficoltà a compararci con quanto accade in un civilissimo Paese anglosassone, negli Stati Uniti.

finalità di controllo della spesa dei presidi farmaceutici, è già prevista la necessità di un controllo dei livelli di appropriatezza

possa stabilire linee guida in cui vi sia un'uniformità di immissione nel mercato sul piano della qualità e dell'appropriatezza dei presidi farmaceutici, non facciamo altro che ribadire quanto il Governo si è già impegnato a fare con le Regioni. Riteniamo

ha fallito il Governo e ha fallito la civiltà di questo Paese nei confronti di oltre 4 milioni di italiani. Signora Presidente, colleghi, questa mozione ci porta ad affrontare un tema delicato che riguarda una malattia che coinvolge purtroppo moltissimi cittadini. Il diabete è una malattia di interesse sociale per la sua alta prevalenza nella popolazione, per il continuo aumento di nuovi casi e per i costi sanitari e sociali che essa provoca. L'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, parla da tempo di «pandemia diabete». Diventa, quindi, indispensabile una strategia di lotta alla malattia che coinvolga tutti gli attori interessati, con l'unico obiettivo di aumentare la consapevolezza generale della dimensione del problema e quindi la possibilità di limitarne l'impatto negativo. I dati statistici in nostro possesso hanno dimostrato e dimostrano che negli ultimi anni, grazie alle terapie e al tipo di impatto utilizzato, nel nostro Paese l'aspettativa

Un ulteriore studio recentemente eseguito ha evidenziato che il 38 per cento dell'eccesso di costo della cura dei diabetici è utilizzato per la cura delle complicanze a lungo termine del diabete, in primo luogo la cardiopatia ischemica e l'insufficienza renale cronica terminale, che sono tra le conseguenze principali di questa malattia. Le conclusioni sono state che il costo medio di un paziente diabetico di tipo 2 in Italia è oggi

Sono spese alte, che verrebbero giustificate se si raggiungesse un obiettivo, ma che debbono essere assolutamente razionalizzate alla luce anche dell'aumentata prevalenza della malattia, che oggi si attesta, come è stato ricordato, tra il 4 e il 5 per cento della popolazione e coinvolge circa 4 milioni di cittadini, considerando anche il diabete giovanile che, purtroppo, è in continua crescita. Dunque, la prevedibile espansione della richiesta sanitaria va di pari passo con una assoluta necessità di contenimento dei costi e di razionalizzazione delle risorse. Diventa quindi indispensabile documentare non solo la quantità delle prestazioni erogate, ma anche il loro contenuto e impatto sullo stato di salute dei cittadini. Altrettanto importante è una giusta collocazione dell'assistenza diabetologica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale affinché la realtà assistenziale per il diabete nel nostro Paese sia efficace ed efficiente. Il modello assistenziale in Italia è oggi un buon modello, che però, rispetto a quello che viene posto in essere in altri Paesi, ha bisogno di un aggiornamento e di una rimodulazione. Tuttavia, come rilevato nella mozione, molto può essere e deve essere ancora fatto per dare risposte più valide, efficaci ed anche più aggiornate a chi soffre di questa insidiosa patologia e soprattutto per contenere contemporaneamente gli elevati costi sociali messi in evidenza. Di questo impegno la politica deve farsi carico e, in riferimento a quanto evidenziato dalla mozione, tale impegno deve tradursi in collaborazione e interazione tra le istituzioni per valutare e verificare le modalità migliori per garantire

razionalizzazione rispetto alle necessità dell'individuo. E ancora, signora Presidente, bisogna intervenire, attraverso documenti tecnici ed etici, in sostegno alla gestione, il che vuol dire anche istituire sistemi di certificazione di qualità delle imprese che intendano concorrere alla fornitura dei presidi e redigere appositi tariffari di riferimento per la fornitura di tali presidi, al fine di garantire la qualità dei dispositivi e l'eguaglianza nella erogazione dei dispositivi e delle cure: una erogazione che sia distribuita in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale. Alla luce di queste considerazioni, annunciamo il voto favorevole su questa mozione. Grazie innanzitutto credo sia doveroso ringraziare ancora una volta la senatrice Baio e tutti i componenti della Commissione sanità che hanno sottoscritto questa mozione, a partire dal presidente Tomassini, per aver riportato per l'ennesima volta sotto i riflettori e all'attenzione di quest'Aula il problema del diabete. In realtà è già successo, com'è stato ricordato da molti colleghi. Mi riferisco sempre ad una mozione di che faceva seguito ad un'interrogazione. Ciò vuol dire che il problema esiste e che è estremamente diffuso sul territorio nazionale. Quei 5 milioni di diabetici conclamati e ormai censiti sul territorio nazionale

La mozione che ci accingiamo ad approvare unitariamente questa mattina ha il significato di voler riportare in auge questo tipo di problematica e di volerla sottoporre alla nostra coscienza.

- va da 0,30 a 0,80 centesimi. Sono importi unitari piccoli, ma la discrepanza è estremamente ampia e la forbice non è sicuramente compatibile

meglio questa indicazione - che la razionalizzazione che dovrà avvenire nello scambio con le Regioni non porti solo ed esclusivamente a un vantaggio economico, ma possa davvero tradursi in una rispondenza precisa ai bisogni dei diabetici. Sarebbe troppo facile riuscire a finalizzare solo dal punto di vista economico, perché cioè con gli oltre 5-6 milioni di diabetici, riuscire a risparmiare pochi centesimi su ogni fornitura vuol dire davvero riuscire a risparmiare parecchi milioni di euro. Questo è sicuramente un obiettivo. L'ottimizzazione delle risorse deve essere assolutamente perseguita, ma non dimentichiamo che deve avvenire solo ed esclusivamente dopo aver avuto la certezza prima ancora che dal punto di vista economico, dal punto di vista qualitativo la fornitura dei presidi ai diabetici sia veramente ottimale e garantita uniformemente

Presidente. Signor Ministro, io la conosco come uomo pratico e spero che le poche parole con cui ha esaurito l'argomento "diabete" significhino, in realtà, una sua precisa presa in carico, nei fatti, dei tre importanti punti con cui il Parlamento sta impegnando il Governo. Ricordo che il Parlamento è la massima espressione della sovranità del popolo italiano. italiano. Il diabete, è stato ricordato anche dagli altri colleghi, è una malattia diffusa, che interessa tutte le età: i giovani, che erano qua prima,

una è quella della diagnosi precoce, dei controlli ambulatoriali nei centri antidiabetici che devono essere più diffusi in Italia e la seconda è il controllo costante della glicemia che avviene attraverso l'autocontrollo del paziente

risparmiando su un'amputazione distribuiamo gratis dispositivi e striscette a decine e decine di pazienti. Allora, voglio ricordare, signor Ministro, che il diabete diventa paradigmatico di due grandi questioni che interessano tutta la sanità nazionale,

La prevenzione e l'autocontrollo non si fanno e le complicanze aumentano. Non a caso, le complicanze sono più frequenti ovviamente nei ceti più bassi della popolazione e queste si riverberano come interventi e ricoveri sul Servizio sanitario nazionale diventando un costo in eccesso che potremmo risparmiare

in sanità sono assolutamente una sciagura perché non si parla di saponette, ma di presidi sanitari e la qualità certificata in questo campo non è un'opzione. Per fortuna, alcune gare al massimo ribasso, è stato ricordato, sono state revocate per la protesta vivace da parte delle associazioni dei pazienti

partito - ma anche dei dispositivi, se vogliamo incentivare l'autocontrollo perché non tutti i pazienti si trovano bene con lo stesso dispositivo e noi dobbiamo garantire davvero l'uguaglianza e l'accesso pieno ai dispositivi e alle cure a tutti. tutti. Concludendo, ben venga questa mozione che tende ad affrontare la questione dell'accesso ai presidi e delle garanzie della loro qualità e disponibilità nel rispetto del diritto di cura del malato. È una mozione su cui il Partito Democratico si esprimerà con voto favorevole sperando che lei, signor Ministro, e il Governo prendiate davvero in carico fino in fondo i punti che questa mozione esprime.

*(PdL)*. Signor Presidente, illustri colleghi, signor Ministro, «(...) Dobbiamo tutti riconoscere che «oggi si fa ancora più necessaria e indispensabile la riaffermazione della centralità della persona umana, perché il nostro contesto storico sembra spesso spingere a considerare la salute come prodotto e il malato come un cliente. E, di conseguenza, la sanità come un ambito del mercato, regolato da analoghe leggi Dionigi Tettamanzi ha pronunciato qualche giorno fa a Milano in occasione della festa del perdono presso il Policlinico; sono parole di una profondità enorme, che rilanciano uno dei temi centrali del dibattito nell'ambito della sanità. Appropriatezza, efficacia, qualità, affidabilità sono parametri evocati sempre più spesso, soprattutto nell'ambito della politica di programmazione, e lo sforzo del legislatore e dell'amministratore, al livello centrale e regionale, è tutto orientato a coniugare questi principi con il governo della spesa, con la economicità. Il tutto di quei principi fondamentali che, ministro Fazio, io desidero ricordare, perché rappresentano punto essenziale, pietre miliari che nello nello schema di piano sanitario nazionale lei ha riproposto in modo assolutamente opportuno come patrimonio della sanità del nostro Paese. Mi riferisco ai principi di universalità, di solidarietà e di equità.

nel contemperare i principi di appropriatezza e di efficacia delle prestazioni erogate con il principio di economicità. Indubbiamente una partita importante nella politica sanitaria - lo sappiamo bene, sappiamo quanto il Governo ed anche le Regioni siano impegnate su questo fronte - si svolge sul versante della prevenzione. Sappiamo benissimo come, nell'ambito della patologia diabetica, il problema della prevenzione sia fondamentale non soltanto per la diagnosi precoce della patologia stessa ma anche per il controllo delle complicanze. L'automonitoraggio glicemico è pertanto una componente indispensabile della gestione della malattia diabetica sia per raggiungere gli obiettivi gli obiettivi di terapia sia per quanto attiene alla necessità di ridurre il rischio determinato da ipoglicemie gravi. È essenziale quindi che il paziente effettui l'autocontrollo con correttezza, continuità e assiduità. A tal di ricordare, come è stato già detto, che il 40 per cento della popolazione diabetica in Italia non effettua alcun tipo di controllo. I sistemi per l'autocontrollo glicemico oggi disponibili sono differenti tra loro, e lo sono non soltanto per il livello di accuratezza e precisione del dato diagnostico, diagnostico, che è un aspetto fondamentale, ma anche per le caratteristiche che ne favoriscono il corretto utilizzo da parte della persona diabetica, adattandosi alle peculiarità di ciascuno a seconda del tipo di diabete, del tipo di terapia, dello stile di vita, del tipo di lavoro, della abilità o disabilità, delle tecnologie, degli aspetti psicologici. Insomma, il dispositivo il dispositivo per la misurazione del diabete diventa addirittura una sorta di elemento sul quale si sviluppa un rapporto empatico tra il paziente e il dispositivo stesso, perché gli aspetti riferiti alla manualità, alla gestione dei dati e alla sicurezza sono fondamentali. Inoltre, va ricordato che questo è un settore dove la ricerca e l'innovazione tecnologica permettono di mettere a disposizione del paziente e del sistema una serie di risultati straordinari che consentono il miglioramento, la maggiore precisione del dato di esame. Inoltre, una scelta del dispositivo medico personalizzata ed appropriata rappresenta un aspetto fondamentale, perché migliora il rapporto costo-beneficio dell'autocontrollo.

determinano una ferita sul percorso difficile che si svolge sul versante della prevenzione ed espongono inevitabilmente ad un pregiudizio per i profili di tutela della salute pubblica.

non hanno sortito alcun buon risultato sotto il profilo del contenimento della spesa, delle procedure amministrative e neanche della qualità del prodotto che si intendeva offrire al paziente. È dunque necessario che, com'è previsto nella mozione, venga lasciata impregiudicata al medico diabetologo ed al paziente la possibilità di di accedere al dispositivo medico migliore per quel determinato paziente. Bisogna pertanto lasciare impregiudicato il principio della personalizzazione del dispositivo medico come presupposto che garantisce la *compliance*. Parimenti, è necessario compiere un passo in avanti sul versante del tariffario nazionale di riferimento, che deve essere costruito sulla base di un'attenta valutazione analitica dei meccanismi di formazione del prezzo di questi prodotti e dei criteri di rimborsabilità, che è auspicabile siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Relativamente a questo aspetto, è indubbiamente apprezzabile, signor Ministro, la tempestività con la quale ha voluto affidare al Parlamento l'Atto del Governo n. 338, relativo alla ricostituzione della Commissione per i dispositivi medici in ambito ministeriale. Vi è poi la necessità di misurare il sistema di utilizzo dei prodotti, al fine di contrastare gli sprechi, spesso correlati a prescrizioni inappropriate o compiere un passo in avanti sul versante dell'educazione terapeutica del paziente, per ridurre progressivamente quella percentuale del 40 un modello distributivo adeguato alle esigenze del paziente, che non generi costi sociali indotti, dovuti anche al tempo e agli spostamenti necessari per il ritiro del presidio

il settore dei presidi e dei dispositivi medici in generale presenta un forte tasso di innovazione tecnologica ed un'enorme potenzialità di sviluppo, che è molto importante. Creare regole che non deprimano questo mercato, ma lo incentivino, vuol dire premiare la ricerca e l'innovazione, che generano qualità: questa indubbiamente ha un costo, che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della disciplina delle gare, le quali non possono essere pilotate soltanto dal criterio del massimo ribasso. Sulla base di questi presupposti, ma anche con questi auspici e con questa diffusa condivisione, a nome del Popolo della Libertà dichiaro in modo convinto l'adesione ed il sostegno a questa mozione.

intervenuto tra i Gruppi, la discussione della mozione sulla diagnosi e la cura del tumore alla mammella è rinviata ad oggi pomeriggio,

quelli che intervengono sull'ordine del giorno a fine seduta hanno il diritto di poterlo fare con tranquillità. Quindi, chi vuole esca, e chi resta abbia un atteggiamento di sostanziale silenzio. *(IdV)*. Vorrei ricordare all'Assemblea che oggi è il secondo giorno di sciopero della fame e del sonno delle agenti della polizia penitenziaria femminile del carcere di Rebibbia; sciopero indetto, come dicevo ieri, per denunciare le gravi carenze di personale. Queste donne meritano la nostra attenzione perché, pur volendo denunciare una situazione davvero insostenibile, hanno deciso comunque di garantire i turni di lavoro, nel rispetto dei diritti delle detenute. Vorrei invitare tutti i colleghi a dare la propria solidarietà alle agenti e soprattutto invitare il Governo a recarsi in carcere a recarsi in carcere per ascoltare le richieste delle agenti e a fornire davvero delle risposte risolutive all'incresciosa situazione; vedo che c'è qualche membro del Governo, e spero siano attenti a questa nostra richiesta.

Il sottosegretario Giovanardi è presente e quindi la sua richiesta di una attenzione da parte del Governo ed eventualmente di un incontro con il personale femminile della polizia penitenziaria è stato recepita: il Governo poi

i *crack* finanziari che avvengono in questo Paese mentre le autorità vigilanti non si sa che fanno.

il problema di un'omessa vigilanza della CONSOB, ma c'è anche un profilo di riciclaggio di denaro sporco da parte di alcune banche, come lo sportello romano della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, la Barclays Bank e altre banche che i magistrati e la Guardia di finanza stanno cercando di individuare. Vede, signor Presidente, ritorno sempre su questo argomento perché non bisogna scherzare con il risparmio,

di una CONSOB che invece di perseguire banchieri e manipolatori del mercato ha chiuso tutti e due gli occhi sulle malefatte dei Tanzi di turno, impiegando risorse ed energie per inseguire teoremi su presunte manipolazioni del mercato a carico di chi denunciava i potentati economici con i quali l'ex presidente Cardia andava a braccetto, in una vera e propria caccia alle streghe. quest'ultimo *crack* non ci sono dubbi. Nel comunicato congiunto CONSOB-Bankitalia dell'11 gennaio venne segnalata al mercato e ai risparmiatori la liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana impresa di investimento di diritto francese, in relazione ad alcune irregolarità. Già questo configura una responsabilità oggettiva di chi non ha vigilato, soprattutto la CONSOB. Per questo, signor Presidente, non c'è nessuna persecuzione. Il signor Cardia ritiene che le nostre denunce siano persecutorie. Non è vero: su omissioni lampanti e manifeste, delle quali dovrà rispondere lui e tutti gli altri della CONSOB, non faccia la vittima, scambiando per persecuzione la sacrosanta tutela - quella sì accanita - dei diritti dei risparmiatori e delle famiglie truffate